signori rappresentanti del Governo, colleghi senatori, la 5a Commissione ha concluso questa notte i suoi lavori senza votare il mandato ai relatori. È per questo che dovete accontentarvi di me anziché della relatrice Zanoni. Sulla base di un *gentlemen agreement* (proposto, per la verità, da una *lady*, cioè dalla senatrice Comaroli, e accettato da tutti i Gruppi), le opposizioni hanno in tal modo rinunciato all'illustrazione, alla discussione e alla votazione degli emendamenti presentati; più di 200. Posto che era evidente che, da parte della maggioranza e del Governo, essendo il provvedimento in terza lettura, l'orientamento sarebbe stato quello di chiedere alla Commissione di respingere tutti gli emendamenti, la Commissione ha ritenuto, quindi, più utile concentrarsi sul confronto su un pacchetto, comunque nutrito, di ordini del giorno, sui quali si è discusso con il Governo. Salvo pochi ordini del giorno che non sono stati accolti, il Governo ha accolto tutti gli ordini del giorno che lo impegnavano ad agire sul piano amministrativo in attuazione di normative già in vigore, di legislazione vigente. Sono stati, invece, accolti come raccomandazione, salvo alcune eccezioni, gli ordini del giorno che comportavano l'impegno a promuovere innovazioni legislative. È evidente che erano impegni che il Governo non poteva assumere, data la congiuntura nella quale ci troviamo, cioè alla fine della legislatura. Per riassumere ai colleghi i contorni del testo che abbiamo al nostro esame, che è stato notevolmente modificato dalla Camera dei deputati, potremmo dire con una battuta, se me la consentite la mia stazza mi fa pensare a queste cose - che il disegno di legge di bilancio è entrato snello in Consiglio dei ministri - così ha detto il Presidente del Consiglio è uscito sovrappeso da Palazzo Chigi (perché già nella fase del dibattito in seno al Governo è cresciuto), è uscito moderatamente obeso dal Senato e, invece, gravemente obeso da Montecitorio. Questa è una prima considerazione di carattere estetico superficiale. Se andiamo un po' più alla sostanza, le cose sono in parte diverse. Lo scheletro della manovra è rimasto inalterato, così come, naturalmente, i saldi. La lettura della Camera dei deputati ha portato in dote risorse aggiuntive in maniera significativa, sia perché ha potuto utilizzare risorse messe in campo dal decreto fiscale - che non era ancora in vigore durante l'esame in Senato - sia perché sono state introdotte misure di potenziamento della lotta all'evasione fiscale, in particolare nel settore dei petroli. C'è stata l'importante misura del riordino e potenziamento delle agenzie fiscali che va in questa direzione, tra l'altro anche a supporto di una delle più una delle più importanti innovazioni di questo disegno di legge di bilancio: la fatturazione elettronica. È stata poi riformulata e potenziata la cosiddetta *web tax*,

di bambini o comunque di figli, in Senato (anche se poi ha visto la luce alla Camera dei deputati) è stato il riordino del pacchetto di misure a favore della

concreto alle famiglie ma si inserisce anche nella filiera dell'avvicinamento dei giovani al lavoro. L'altro elemento di potenziamento delle detrazioni fiscali riguarda il pacchetto ecobonus e sismabonus che è stato significativamente potenziato. Veniamo alla parte spesa. C'è una parte significativa di norme di spesa che presentano anche alcune criticità, sulle quali credo sia opportuno che il Senato ragioni. C'è una sistemazione dalla spesa Regioni, Province, Comuni e autonomie speciali, per circa 500 milioni; c'è un potenziamento dell'Ape sociale e poi - questo

in particolare nel comparto scuola, università e ricerca. Con questo ho concluso l'illustrazione dei contenuti essenziali. Mi permetto di fare due considerazioni, da Presidente della Commissione, non da relatore: lo dico allo stimato collega Calderoli. La prima. È del tutto evidente che la riforma della legge di bilancio della legge di bilancio che abbiamo approvato due anni fa stenta a entrare in vigore. Abbiamo introdotto significative innovazioni che dovevano mirare anche ad alcuni obiettivi; il risultato di questo lavoro ci consegna una situazione problematica, sulla quale credo che il prossimo Parlamento dovrà riflettere e ragionare. In particolare, il vaglio parlamentare sostanzialmente ancora ignora la struttura complessiva della spesa, la dà per scontata, la dà per acquisita, se ne occupa il Governo.

richiamato - ma il dibattito parlamentare e la pressione che avvengono attorno alle due Commissioni bilancio di Senato e Camera, naturalmente con le dinamiche diverse che tradizionalmente ci sono in questi due rami del Parlamento, si concentrano su una massa di interventi al margine, tutti di aumento di spesa corrente o per lo meno prevalentemente di aumento di spesa corrente, spesso permanente e strutturale. Io credo che questo ci consegni un problema per il Paese e per il Parlamento, ossia come recuperare - fatemelo dire - quello spirito einaudiano del dibattito all'interno della Costituente nel quale questo grande Padre della nostra Costituzione - ieri è stato giustamente ricordato l'anniversario dell'approvazione della Carta temeva che questa deriva del Parlamento capovolgesse il senso del parlamentarismo originario. Il Parlamento nasce come luogo di rappresentanza dei contribuenti e di sorveglianza dei contribuenti rispetto alla volontà di spesa del re, cioè del Governo. Invece, rischia di trasformarsi in un'Assemblea che chiede spesa al Governo; in un'Assemblea - passatemi il termine un po' forte - di sudditi che chiedono al sovrano più spesa. Non a caso, Einaudi voleva evitare l'emendabilità delle leggi di spesa in Parlamento. Questa proposta non fu accolta e, in suo luogo, fu introdotto l'articolo 81, a presidio del quale ci sono le nostre Commissioni, ma - com'è noto - è un presidio che fa fatica a sostenere. Io credo che questo sia un problema che questa legislatura lascia in eredità alla prossima. Chiunque sarà al Governo avrà a che fare con questo problema. Ciò tanto più è l'ultima considerazione che faccio, colleghi - che questa abitudine alla pressione sulla spesa, a conquistare spazi di spesa (spesso spesa corrente strutturale e permanente, ognuna delle quali ha mille giustificazioni, ma nell'insieme dipingono un quadro difficilmente sostenibile), rischia di collidere con la congiuntura di carattere economico nella quale siamo, che è una congiuntura per fortuna positiva. Abbiamo spazi di manovra più ampi rispetto a quelli di inizio legislatura, ma proprio questo ci deve indurre a utilizzare una parte significativa del dividendo della crescita in termini di margini di finanza pubblica

con i ringraziamenti del caso, che riguardano non solo questa sessione di bilancio, ma un po' l'intera legislatura. La 5a Commissione - che so essere la Commissione più «amata» dai colleghi senatori, perché è la più «popolare», quella che è costretta tante volte a dire dei «no» molte volte sgradevoli ha tenuto 858 sedute in questa legislatura: un *record* ineguagliabile da parte di qualunque altra Commissione. Ringrazio il Senato, innanzitutto il Gruppo del PD che mi ha proposto, i Gruppi della maggioranza che mi hanno eletto, e poi tutti i senatori e i Gruppi dell'opposizione, con i quali ho collaborato, per l'onore che mi è stata fatto di presiedere questa importante Commissione, in uno spirito che è stato sempre di leale confronto e di collaborazione - ripeto - anche con i Gruppi dell'opposizione. Ringrazio tutti i senatori per la comprensione nei confronti dei nostri rilievi e dei nostri richiami, che spesso sono sgradevoli. Io dico che la 5a Commissione ha il compito di presidiare il principio di realtà, mentre spesso le altre sono molto attratte dal principio di piacere (tutte le cose che si vorrebbero fare) e poi c'è il richiamo al principio di realtà, che spesso non è popolare né gradevole, ma è doveroso.

della riforma costituzionale ed è fortunatamente sopravvissuta al naufragio della riforma stessa; credo sia un tema da recuperare se vogliamo riprendere quello spirito einaudiano di cui parlavo prima. Ringrazio poi il Servizio del bilancio, in particolare il dottor Loiero e tutti i suoi collaboratori, per il lavoro continuo e assiduo di documentazione, di straordinaria professionalità*.* ringrazio la segreteria della Commissione, con la quale lavoriamo gomito a gomito quotidianamente, diretta in modo eccellente dalla dottoressa Piccardi,

quindi il suo invito è un monito che va raccolto e la ringrazio per questo. Onorevoli colleghi, in relazione a quanto riferito dal senatore Tonini, il disegno di legge n. 2960-B, non essendosi concluso l'esame in Commissione, sarà discusso nel testo trasmesso dalla Camera

Signor Presidente, innanzitutto vorrei farle i migliori auguri perché, anche se in pochi lo sanno, oggi dovrebbe essere il suo compleanno.

i nostri nonni erano talmente impressionati dalla guerra che hanno cercato di rivelarmi il 1° gennaio 1945, pur essendo nato il 23 dicembre 1944, in realtà prematuro. Scusate di questo siparietto personale, ma mi ci ha spinto il senatore Calderoli. concluso l'esame in Commissione, però mi è piaciuto moltissimo il paragone rispetto alle manovre che nascono magre e che finiscono grasse, perché si rappresenta anche in quest'Aula:

Signor Presidente, onorevoli senatori, a nome del Governo, autorizzata dal Consiglio dei ministri, pongo la questione di fiducia sull'approvazione, senza emendamenti, subemendamenti o articoli aggiuntivi, dell'articolo 1 del disegno di legge n. 2960-B (Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2018 e bilancio pluriennale per il triennio 2018-2020), nel testo approvato dalla Camera La Presidenza prende atto dell'apposizione della questione di fiducia sull'approvazione dell'articolo 1 del disegno di legge n. 2960-B, nel testo identico a quello approvato dalla Camera dei deputati. Convoco pertanto la Conferenza dei Capigruppo per organizzare il relativo dibattito. La seduta è sospesa.

parlamentari ha proceduto all'organizzazione dei lavori sulla questione di fiducia posta dal Governo sull'articolo 1 del disegno di legge di bilancio per l'anno finanziario 2018, nel testo approvato dalla Camera dei deputati. Per la discussione sulla fiducia sono stati ripartiti trenta minuti sulla base di specifiche richieste dei Gruppi. Seguiranno, quindi, le dichiarazioni di voto. La chiama avrà inizio orientativamente alle ore 11. Dopo il voto di fiducia si passerà alla votazione dei restanti articoli e dei relativi emendamenti, nonché alla votazione finale con procedimento elettronico del disegno di legge.

ha finito di occuparsi delle banche di papà e di tutti i numerosi conflitti d'interesse che ne hanno caratterizzato l'operato. E non mi limito a richiamare quello clamoroso della Boschi, di Renzi e del PD per Banca Etruria o per Monte dei Paschi di Siena. Sono stati in grado di offuscare le famigerate leggi *ad personam* per l'ex senatore Berlusconi, oggi dipinto dai suoi valvassini come una sorta di redivivo santo moralizzatore: i suoi fidi Brunetta e Gasparri oggi si mostrano agli italiani come fantomatici uomini di Stato, dopo aver fatto a pezzi il Paese quando sono stati al Governo. Di certo, sottovalutano la memoria degli elettori, che ancora oggi stanno pagando l'incapacità e la malafede di una classe politica che, dal PD a Forza Italia, ha pensato più alle minigonne e ai bancomat che al futuro dei nostri ragazzi. Del resto, chi può dimenticare i consigli affabili di Berlusconi, che da Presidente del Consiglio invitava le ragazze italiane non già a studiare, ma a scegliersi un marito facoltoso come suo figlio? Oggi, in questa maggioranza in fuga, come non possiamo ricordare lo scandalo TAP (Trans Adriatic Pipeline) e il farneticante tentativo del ministro Calenda, in quest'ultimo fine settimana, di far approvare in Commissione la vergognosa militarizzazione di una delle più belle aree del nostro Paese? al meraviglioso Salento, in cui si è pensato bene di espiantare migliaia di ulivi secolari per fare spazio a un gasdotto inutile e pericoloso. proprio del ministro Calenda, quello che utilizza il proprio Ministero per attaccare ingiustamente Virginia Raggi e coprire gli indegni affari che la sua area politica di appartenenza ha compiuto negli ultimi anni sulla pelle dei cittadini di Roma. Quello stesso ministro Calenda che nei giorni scorsi, in occasione del pericoloso incidente verificatosi in un impianto di distribuzione di gas in Austria, ha difeso la presunta importanza strategica della realizzazione del gasdotto TAP nel cuore delle bellezze naturali della mia amata Puglia. emendamento, soprattutto dopo le proteste del Movimento 5 Stelle, è stato dichiarato inammissibile. Per questo ringrazio il collega Boccia, che, anche in quest'occasione, magari con maggiore fortuna, ha favorito le ragioni della pace, al pari dell'ipotizzato utilizzo dei famigerati F35 F35 con cui suggeriva di spengere gli incendi, confondendo aerei da guerra con innocui Canadair. Ma va bene così, in fondo anche Boccia fa parte del PD. Nonostante il fallimento dell'iniziativa di Calenda, resta l'arroganza di un gesto che, ancora una volta, ha messo in luce gli scandalosi conflitti d'interesse che avvolgono il Governo. Calenda opera da mesi come un Ministro della TAP. Del resto, il nuovo capo di gabinetto, come pubblicato da «L'Espresso», è un uomo TAP: è clamorosamente un uomo del consorzio TAP. Insomma, il Ministero per lo sviluppo economico è oggi gestito da un'azienda privata

sono sempre ai loro posti, mentre i giovani del nostro Paese continuano a non trovare lavoro, affondando nella precarietà, come accade per i ricercatori del CNR di Bari. E, nel frattempo, questo PD ha affossato definitivamente la possibilità di abolire i vitalizi. La verità

L'antico vizietto di chiudersi nel Palazzo e di rendere complicato per i cittadini poter accedere liberamente a un'equa e uguale informazione - com'è accaduto qualche giorno fa in Commissione di vigilanza RAI, dove tutti i colleghi hanno votato contro la nostra richiesta di trasmettere i lavori

è palese, evidente e - a mio parere - scandalosa. Mi auguro che i cittadini italiani facciano presto giustizia, restituendo a questa meravigliosa Nazione la possibilità di riprendere a sognare un futuro migliore per tutti: per come la penso io, un futuro a cinque stelle.

Presidente, onorevoli colleghi, il tempo a disposizione è pochissimo, per cui faccio subito gli auguri di buon Natale e buon anno a tutti voi e alle vostre famiglie.

le imprese che non ci sono state, con livelli di tassazione che sono i più alti di Europa; alla crescita a livello di prefisso telefonico

modo, in questo disegno di legge di bilancio abbiamo la definizione di chi si prende cura: finalmente lo Stato inizierà a prendersi cura di chi si prende cura, e questo è un già un punto di arrivo. Abbiamo istituito un fondo che - lo voglio specificare - è vincolato, non si fanno divisioni: il fondo è vincolato a eventuali disegni di legge che saranno fatti per loro.

se solo riusciste a dare qualche giorno a questa legislatura scalcagnata, potremmo sicuramente portare a casa due risultati importantissimi. Il primo

Purtroppo, esistono problemi che lascio e - ne sono consapevole - non si potranno risolvere sicuramente in questa legislatura, ma che certamente sono degni di un cenno. Abbiamo insegnanti di sostegno impreparati; una scuola che non gestisce nella maniera più assoluta

E soprattutto resta il *vulnus* per la scuola: abbiamo introdotto l'alternanza scuola-lavoro, ma non esiste una sola parola scritta su come si debbano gestire i ragazzi disabili in questo caso.

Signor Presidente, molto probabilmente questa è l'ultima volta che parlo in quest'Aula e soprattutto che intervengo in discussione generale per una legge di bilancio.

al bene pubblico. Al contrario, sono orgogliosa di appartenere a un Movimento che ha sempre lavorato solo ed esclusivamente in funzione del bene di tutti i cittadini, senza voler tutelare una sola parte a discapito di altre, senza voler garantire prevalenze o privilegi ad alcuno. Sono orgogliosa del Movimento al quale appartengo e di come i miei colleghi hanno lavorato e si sono spesi fino all'ultimo in questa legge di bilancio, sia al Senato che alla Camera, partecipando alle numerose e lunghissime sedute di Commissione. Doveva essere salvaguardata la disorganizzazione di un Governo e di una maggioranza che non sono stati in grado neppure di garantire bene le coperture degli emendamenti che voleva portare a casa, continua disorganizzazione e competizione tra i Gruppi politici che sono all'interno di questa Aula, per mettersi d'accordo e strappare il contentino da garantire al proprio territorio o alla propria *lobby*, che li ha portati qui dentro e li sostiene per la prossima campagna elettorale. Nonostante le accuse fatte alla Banca d'Italia e nonostante Renzi, in questi giorni, non abbia fatto altro che tentare di discolparsi la vicenda grave di Banca Etruria e le collusioni emerse all'interno di una Commissione di inchiesta che è stata avviata - quella sì,

una misura che, con coerenza decisionale, era necessario inserire: ovvero, tassare il bilancio della Banca d'Italia con una minima percentuale, pari all'uno per cento al netto delle voci rettificative del passivo, come come è stato proposto nel disegno di legge che ho depositato e nell'emendamento dal quale era tratto. la tassa applicata sul totale della attività del bilancio della Banca d'Italia avrebbe segnato una inversione di tendenza rispetto al fare debito, che prima prima veniva ben citato, e avrebbe aumentato il *plafond* di questo bilancio con più di sette miliardiche, seppure non sono di spesa corrente, sono una ingente cifra. Non si sarebbe corso il rischio di ledere l'indipendenza finanziaria e istituzionale della Banca d'Italia, in quanto si stabilisce che

competente in modo esclusivo rispetto agli altri Stati ed è legittimato a legiferare in materia fiscale. Concludo, dicendo che molti emendamenti proposti dal nostro Movimento, e sono tutti a fini di bene pubblico. Signor Presidente, intervengo su un tema molto specifico. In particolare, intervengo sul comma 568, lettera

l'importo delle opere che i concessionari autostradali possono fare senza gare d'appalto. E ciò crea un problema profondo. In 8a Commissione, il presidente Matteoli riuscì, su proposta di tutti i componenti, di tutti i Gruppi, ad avere il contratto di concessione di Autostrade per l'Italia, che noi abbiamo studiato; e abbiamo anche presentato un esposto all'ANAC su questo tema. *(Applausi dal Gruppo M5S)*. il valore di investimento, che è quello che determina la tariffa, è stato sopravvalutato. In particolare, si considera che il valore di investimento, derivante dal computo metrico, è stato scontato, nella convenzione, del 15 per cento, piuttosto

sta per firmare una proroga della concessione e, oltretutto, aumenta il valore di investimento di altri 6,7 miliardi, concedendo poi ad Autostrade per l'Italia una buonuscita di 5,7 miliardi.

2013: un bel regalo di Natale. Adesso il ministro Delrio sta firmando un nuovo atto. Noi pensiamo che i regali di Natale debbano essere fatti ai cittadini, che queste cose siano assolutamente fuori dal mondo, che bisogna fermare un tale scempio e che le concessioni debbano pubbliche. Abbiamo raffrontato la concessione di Autostrade per l'Italia con la concessione di Aeroporti di Roma, essendo il concessionario lo stesso, e cioè la società Atlantia, controllata a sua volta dalla società Edizione srl, il cui amministratore delegato è "stranamente" l'ex amministratore delegato di Telecom Italia Patuano, Queste persone tornano sempre, sono sempre loro. Noi vediamo che nell'ambito del contratto di Aeroporti di Roma c'è trasparenza, perché pubblicato sul sito dell'ENAC mentre sul contratto di Autostrade per l'Italia non c'è trasparenza. Il ministro Delrio non pensi di firmare quella proroga, e soprattutto non pensi di poter scaricare la responsabilità sul funzionario che materialmente firmerà l'atto. Noi vigileremo, anzi porteremo immediatamente le carte all'autorità giudiziaria, e quindi, denunceremo il Ministro dal punto di vista penale se farà questo. Non è pensabile che a fine legislatura si faccia un regalo ai soliti potenti. Quello che vediamo è che si colpiscono sempre le persone normali. Ma, quando si trova uno che ha il potere economico di influenzare la politica, non lo si colpisce mai. Questo è il motivo per il quale non avete più ragione di esistere, né da una parte né soprattutto dall'altra. Quelli poi di una certa parte non hanno proprio ragione, perché non hanno mai difeso gli interessi, anzi sono sempre stati in conflitto di interessi. A sentire ancora oggi Berlusconi parlare di rivoluzione liberale viene veramente da vomitare: lui che ha ucciso

in realtà, viste le condizioni, avevo deciso di non intervenire affatto, ma questa maggioranza e questo Governo non perdono occasione di far capire da che parte stanno, e cioè della parte dei forti.

in una discussione amichevole, il senatore Santini mi ha detto che siamo molto fantasiosi nel dire cose contro il *jobs act*. Questo fa parte di ciò che voi dite, senatore Santini. Le voglio però ricordare una cosa: lei ha praticamente la mia stessa esperienza e chi nasce sindacalista lo è per sempre. Se lo ricordi, perché siffatte nefandezze - naturalmente non lo dico solo a lei, ma a tutti - i lavoratori proprio non le meritano. A questo punto è giusto che questa legislatura finisca, perché è stata veramente pesantissima e una tragedia per chi sul serio vuole rappresentare la parte sana di questo Paese.

Signor Presidente, intervengo sul disegno di legge di bilancio in esame per far presente a tutti, e soprattutto ai cittadini che ci ascoltano da casa, che anche quest'anno, come per gli altri quattro già trascorsi, il Governo e la maggioranza hanno perso l'occasione di dare una visione di futuro all'Italia. Senza provvedimenti strutturali non si creano né fiducia né stabilità, non si traccia quel percorso che serve a tutti per andare nella stessa direzione. Vi abbiamo visto correre e rincorre Ministri e Sottosegretari per far approvare emendamenti, per poter permettere a qualcuno di portare avanti una sua personale campagna elettorale, o per portare soldi a fondazioni e aziende dei soliti amici degli amici. Tutto questo fa male all'Italia e dimostra che non siete credibili. Tanti sono gli errori che avete perpetrato e che si potevano evitare, come la decontribuzione al 50 per cento per imprese che assumono a tutele crescenti. Ci aveva già provato Renzi, bruciando 20 miliardi in tre anni di decontribuzione al 100 sui contributi previdenziali; ma sono stati soldi buttati, considerato che hanno spinto le imprese ad assumere col contratto a tutele crescenti solo per percepire il *bonus*, La decontribuzione ha creato una bolla di nuovi contratti a tutele crescenti, che si è sgonfiata appena Renzi ha ritirato l'incentivo (dal 2016).

Il lavoro stabile non si crea né con le norme come il *jobs act,* né con gli incentivi, ma si crea con gli investimenti produttivi che creano domanda stabile per le imprese e quindi necessità di nuovi posti di lavoro. Ce ne sono tantissimi da fare, sia ordinari come la manutenzione del territorio e nel trasporto pubblico, sia innovativi come la riconversione dell'economia dal fossile alle rinnovabili, o come nel settore del risparmio energetico, e una politica credibile e precisa nello sviluppo reale della banda ultralarga. Se non avremo un Governo che opererà seriamente in questi settori e con continuità, i risultati saranno sempre gli stessi, cioè quelli fallimentari di questo Governo, che va avanti con operazioni a gettone: se mette il gettone, la giostra gira; se non lo mette, la giostra si ferma. proroga dell'ecobonus*.* Da tempo si continua a prorogare l'ecobonus di un solo anno alla volta, anziché stabilizzarlo per almeno cinque anni come ha sempre chiesto il Movimento 5 Stelle. La proroga annuale non permette alle famiglie e alle imprese di progettare e, per le imprese, fare piani a lungo termine vuol dire tutto. Avere una stabilità normativa che consenta di programmare l'investimento è alla base di un'impresa. Con la stabilizzazione dell'ecobonus si sarebbe inoltre potuta creare tantissima nuova occupazione. Questo Governo, invece, ha ridotto l'ecobonus dal 65 al 50 per cento per molte tipologie di interventi e quindi, in parte, ha fatto anche peggio del Governo Renzi. l'attacco alla sanità. Da qui al 2020 è prevista una riduzione degli investimenti destinati alla sanità ed è un dato allarmante, se consideriamo che la maggior parte delle persone

Anche nella legge di bilancio 2018 ci sono tagli diretti e indiretti al fondo sanitario nazionale per miliardi di euro. A pagare il conto sono le fasce più deboli, spesso costrette a rinunciare alle cure a causa delle lunghe liste d'attesa e del costo eccessivo della sanità privata, che cresce. La prospettiva di una sanità di serie A e di serie B si sta concretizzando anno dopo anno. Anche per il 2018 il Governo ha previsto tagli ingenti rispetto alle previsioni iniziali. Le risorse complessive per l'anno prossimo erano state fissate a 114 miliardi di euro, poi, con un decreto ministeriale sono state ridotte di 604 milioni, a cui si aggiunge un'altra riduzione di 94 milioni di euro per l'edilizia sanitaria. Dunque, ricapitolando, non c'è nulla di concreto per combattere la disoccupazione giovanile, per supportare gli enti che si trovano in condizioni di dissesto finanziario a causa della *spending review:* nulla di nulla. Anche in questa occasione, se ci sono state poche cose positive approvate è merito nostro e del nostro lavoro. D'altronde, noi del Movimento 5 Stelle non abbiamo bisogno di ringraziare nessuna *lobby* che ci finanzia le campagne elettorali. Noi agiamo solo per il reale interesse dei cittadini. *(Applausi dal Gruppo M5S)*. Le sole cose positive che leggiamo in questa legge sono quelle che ha fatto approvare il Movimento 5 Stelle, come l'emendamento del collega Vignaroli, con il quale si riconosce un credito d'imposta del 36 per cento alle imprese che acquistano prodotti realizzati con materiali derivati da plastiche miste provenienti dalla raccolta differenziata degli imballaggi o da selezioni di rifiuti urbani residui. del collega Fraccaro: finalmente anche in Italia saranno introdotti quei sistemi con cui un'auto elettrica può cedere energia alla rete, rendendola un sistema intelligente. È un bel modo, questo, di usare le tecnologie. Poi c'è l'emendamento Giordano, che aumenta lo stanziamento del fondo per la cura dei soggetti con disturbo dello spettro autistico di 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2019 e 2020. Insomma, queste sono solo alcune delle proposte che siamo riusciti a far passare - e la differenza, rispetto alle vostre proposte, si vede e si nota - proposte utili e pratiche, che fanno bene ai cittadini e alle imprese, diminuiscono i consumi e gli sprechi e aumentano l'occupazione, creano nuove opportunità e forniscono cure a chi ne ha bisogno. Gentili colleghi, forse questo è il mio ultimo intervento in quest'Aula e, volendo fare una riflessione, devo dire che sicuramente siamo cresciuti qui dentro in esperienza e fuori fuori dal palazzo in numero, a causa di tutte le vostre pessime scelte, che hanno rappresentato per noi delle battaglie condotte al fianco dei cittadini; come quando volevate la privatizzazione dell'acqua, o avete dato il via libera a nuovi inceneritori in Italia, o quando avete tolto i soldi alle persone per darli alle banche, o infine quando addirittura eravate tutti convinti di voler abolire perfino il Senato della Repubblica e noi, assieme al popolo Congratulazioni)*. Insomma, se sta per arrivare un nuovo Governo, il primo Governo dei cittadini, senza *lobby*, è anche un po' grazie a voi, che avete fatto capire a tutti che l'unica soluzione è un Governo a 5 Stelle. In alto i cuori, cittadini!

spiego, dal mio punto di vista, qual è stata la vera storia della *web tax*, come la Camera ha snaturato il provvedimento approvato dal Senato e come in questo modo si rischia di non avere il gettito che viene proposto, stimato e speso.

minuti, utilizzando un linguaggio rigoroso e riferito alla verità dei fatti. Sono passati cinque anni e abbiamo dimenticato che questo Parlamento e questa legislatura sono nati in una fase di crisi profonda del Paese; in una situazione nella quale si raccoglieva il risultato di un Governo

in una profonda crisi economica, sociale, istituzionale e politica;

dovremmo dire che restituiamo il Paese in una condizione veramente diversa tutti i proclami che ancora si sentono e anche le propagande, che anticipano da tempo la campagna elettorale, le quali si dà un'immagine del Paese e delle sue istituzioni ancora più pesante di quella vissuta nella precedente legislatura. Purtroppo, signor Presidente, cari colleghi, così non facciamo onore neppure a noi stessi: lo dico anche a quelli che più di ogni altro usano toni aggressivi. Questa è una legislatura nella quale molti provvedimenti sono stati adottati a larghissima maggioranza, nella quale si sono fatti passi da gigante sul piano dei diritti umani e civili

Basterebbe segnalare alcuni di questi punti per dire che quelle parole e quelle propagande aggressive sono veramente esorbitanti rispetto alla realtà.

che una delle norme - ma è una delle tante - riguarda la bonifica dei poligoni italiani. Oggi abbiamo una procedura chiara, che interviene a bonificare, in caso di esercitazione, entro centottanta giorni tutti i poligoni italiani, a salvaguardia della salute degli operatori della difesa

credo che andiamo verso una campagna elettorale molto difficile e complicata, che non darà al Paese neppure certezza di Governo. E chi pensa che un arretramento dello schieramento avanzato possa premiare qualcuna delle sue componenti certamente sbaglia. Se qualcuno pensa che l'unità che andrebbe trovata nell'ambito dello schieramento democratico invece vada evitata, credo non faccia credo non faccia il bene del Paese e neppure il bene della nostra democrazia. Penso che dovremmo riflettere, in queste ore e giorni, su questo argomento e lavorare di più e meglio. Porgo gli auguri a lei, signor Presidente, a tutta l'Assemblea e a tutti i funzionari che ci hanno assistito con grande pazienza in questo lavoro, agli assistenti parlamentari, che spesso si sono dovuti frapporre,

Auguro a tutti buone feste e auguro anche a tutti di poterci ritrovare, se non qui comunque nella storia politica di questo Paese, a difendere le nostre convinzioni con rispetto verso gli altri. Governo, colleghe e colleghi, questa è l'ultima legge di bilancio di questo Governo e l'ultima fiducia di una sequenza innumerevole di voti di fiducia ai quali abbiamo sempre risposto con un no convinto. Non certo un no per parte presa, non rientra infatti nel nostro modo di lavorare, ma per la totale assenza di un disegno strategico capace di dare risposte adeguate ai problemi dei nostri cittadini, ai problemi e alle difficoltà che sono sotto gli occhi di noi tutti, forse non sotto i vostri. allora quanto già espresso, evidente anche in questa fase: una chiara e netta fotografia di una maggioranza che in modo fallimentare maschera tutte le debolezze delle tensioni interne, della difficoltà di convergere in un disegno di riforme strutturali ed incisive, necessarie ed inderogabili. forte l'assenza di una visione strategica di medio e lungo termine, da noi sempre auspicata. Ed allora se parte di quegli interventi da noi richiesti in prima lettura al Senato non hanno trovato risposta, forse perché presentati dall'opposizione e quindi non degni di nota, anche se pieni di contenuti, alla Camera, dove la maggioranza è più ampia ed i rischi sono nulli, sono stati ripresi al solo fine di poter dire: «Questo lo abbiamo fatto noi». Infatti, tra l'altro, le risorse sono emerse a iosa, come prima ha detto il Presidente della Commissione bilancio: è stato veramente come espletare una nuova legge di bilancio alla Camera, con una ricchezza, un'opulenza, una quantità di denaro che al Senato purtroppo non era disponibile. Tornando alle proposte, ricordiamo che erano e sono le nostre proposte, proposte di chi ha una visione diametralmente opposta alla vostra e per le quali è innegabile la consistenza, tant'è che poi ne avete fatto uso. Siamo convinti che un rapporto costruttivo nasca dal saper cogliere quanto sa dire chi ha a cuore le nostre famiglie, i nostri giovani, i nostri anziani, questo nostro Paese nel suo complesso, per poter costruire un futuro concreto, un futuro fatto di stabilità, di possibilità di programmare il futuro stesso. molte delle nostre proposte, quindi, sono state portate in seconda lettura, pur di non lasciare spazio alle minoranze. Ma ben venga, lo diciamo convintamente, il vostro passo indietro. A noi non interessa piantare le bandierine, ci interessa il bene del Paese e quindi il risultato. Pensiamo alle risorse per il settore zootecnico praticato nelle zone montane o disagiate, o alla stabilizzazione per la detrazione dei canoni degli alloggi universitari per i fuori sede residenti in zone disagiate o montane, la cui distanza è ridotta a 50 chilometri: un nostro emendamento che abbiamo presentato nel decreto cosiddetto fiscale, un emendamento fortemente

perorata quindi come indispensabile per sollevare donne che, con abnegazione, devono farsi carico spesso - anzi, direi quasi sempre - di un sistema socio-assistenziale carente. Qualcosa è stato fatto, dobbiamo dirlo. Molto è stato ripreso da quanto presentato in prima lettura al Senato, ma troppo resta da fare. Ci si aspettava maggiori risposte e meno proroghe, adatte ad altri provvedimenti, non certo ad una legge di bilancio. Ma la scelta più grave, che riguarda proprio le proroghe, è quella sulla quale non possiamo non puntare il dito; riguarda infatti gli apparecchi del gioco lecito. Mentre anche gli enti locali si sforzano con le poche risorse che hanno di disincentivare le voi prorogate il termine per il rilascio del nulla osta; il tutto con costi sociali enormi, con risvolti sociali che sono gravosi e a volte disastrosi per le famiglie e per i singoli e purtroppo con effetti a lungo termine dannosi. In cambio di che cosa? In cambio di liquidità immediata, in cambio della possibilità di avere risorse fresche che andranno poi disperse negli anni a riparare i danni che tutto ciò comporterà. Noi abbiamo continuato a sollecitare e a chiedere misure che ridiano dignità,

stabili, quelle che noi sicuramente daremo. Noi con l'Italia voterà no a questa fiducia.

chiedo l'autorizzazione a consegnare il mio intervento scritto, nel quale ne vengono enunciate le motivazioni. Colgo l'occasione per augurare a tutti i colleghi a tutti i funzionari del Senato e della mitica Commissione bilancio - e ovviamente di tutta la struttura - un sereno Natale e soprattutto un buon anno. *(Applausi).*

anche noi diamo il nostro contributo a questa legge di bilancio, un contributo importante e determinante perché la nostra

siamo estremamente lieti di aver contribuito a permettere, in questi anni, che il Paese avesse quelle riforme

che si sono quindi eruditi sulle tecniche legislative e parlamentari; di questo ovviamente

tutti i colleghi e i funzionari che in questi anni hanno accompagnato, sotto la guida del presidente Tonini e del presidente Azzollini, il lavoro della Commissione bilancio. È un voto contrario che esprimiamo con rammarico, auspicando che,

la legislatura finisce nello stesso modo in cui varie volte si è contraddistinta in questi anni:

Al netto della propaganda che ogni tanto si è fatta contro le politiche di *austerity*, in realtà si è riconfermata nel tempo. In questa legislatura sono state fatte scelte all'insegna della precarizzazione del mercato del lavoro, dei *bonus*

la capacità produttiva del 27 per cento; il PIL del 6,4 per cento. Ci sono 11 milioni di italiane ed italiani che rinunciano a curarsi perché non possono pagare i *ticket*; 5 milioni di persone vivono in condizioni di povertà assoluta. Tra l'altro, proprio qualche settimana fa, l'ISTAT ci ha detto che metà delle famiglie italiane è a rischio povertà. Questi sono i dati e non si può far finta di nasconderli. Quindi, dopo tutti questi anni della vostra cura di *spot* pubblicitari, l'Italia alla fine si ritrova come un Paese più disuguale, in cui i poveri sono aumentati, c'è più sofferenza sociale e più depressione economica. Avete sbagliato le politiche. Avete privilegiato, nei fatti, regalie fiscali e alle imprese; avete scelto il *bonus* bebè invece che gli asili nido; avete trasformato il mercato del lavoro in un mercato dei lavoratori, i lavori in lavoretti.

bisognava fare. Avete scelto questa formula per due motivi: per una ragione elettoralistica e pubblicitaria e, di fatto, per la scelta ideologica di una politica economica fallimentare. Signor Presidente, colleghi,

di uscita dalla crisi che, a nostro avviso, si è dimostrata completamente sbagliata, e i dati che ho citato prima lo stanno a dimostrare. I 62 miliardi di euro che sono stati a nostro avviso buttati al vento in una politica fatta semplicemente di incentivi a pioggia e di *bonus*,

Le disuguaglianze, lo ribadisco, sono aumentate e non serve a niente un w*elfare* fatto per *spot* e piccoli annunci, come quelli della lotta alla povertà, che poi non hanno sostanza e strutturazione. Noi invece pensiamo che sarebbero state necessarie

allargare l'istruzione nel nostro Paese e investire nella scuola e nella ricerca; abolire i *superticket*; recuperare risorse (cancellando ad esempio il programma degli F-35) e aumentare l'imposizione fiscale su chi più ha e può dare a questo Paese. Pensiamo appunto un intervento che sarebbe stato necessario, ossia non meno tasse per tutti, ma per chi già ne paga tante, e più tasse per chi ha un grande patrimonio. Questi sono gli obiettivi che abbiamo tentato

che il Presidente del Consiglio ha riscoperto i cambiamenti climatici, ma badate bene che per opporsi e fare un piano che

su un processo serio di affrancamento. Invece le scelte, anche in questa politica di bilancio, sono state ancora una volta non solo parziali ma per certi versi addirittura in controtendenza rispetto a scelte di politica energetica.

dalla crisi e di avere una speranza di futuro. Il lavoro è la principale fonte di questa ricchezza: investire nel lavoro, nel w*elfare* e nei diritti è il nostro piano per arrivare alla definizione di un programma vero

Signor Presidente, questa è la ventiquattresima volta che seguo una legge di bilancio. Rispetto agli anni Novanta il contesto è molto più complesso e le risorse a disposizione sono molto meno di una volta. Ciononostante, credo

ossia con la procedura accelerata prevista dall'articolo 104 dello Statuto. Un risultato così, dal 1948 a oggi, non si è mai verificato. Oltre alla competenza sull'energia, siamo riusciti a ottenere l'attribuzione della competenza sui tributi locali e sulla finanza locale. C'è stato un nuovo accordo finanziario che ha responsabilizzato le nostre Province, dove - lo ricordo ai colleghi - ben un miliardo di euro viene versato alle casse dello Stato. In cambio, abbiamo ottenuto la possibilità di programmare meglio i nostri bilanci, contribuendo al risanamento del bilancio statale statale e ottenendo una certezza del diritto e meno interferenze da parte dello Stato. Siamo riusciti anche a sbloccare i fondi dovuti dallo Stato per la Valle d'Aosta e per le nostre due Province, il che consentirà una piena ed efficace politica di bilancio per i

quasi dieci anni, che ha raggiunto il suo culmine durante il Governo Monti, quando vennero adottate misure drastiche contro con le autonomie speciali, con il rischio di minare la base delle stesse. Per questo motivo, abbiamo sostenuto con convinzione prima il Governo Letta, poi, il Governo Renzi e, adesso, il Governo Gentiloni Silveri, che si sono sempre dimostrati sensibili alle esigenze delle nostre autonomie. Vorrei ringraziare, in particolare, il presidente Napolitano, ma anche il Ministro

non solo per la grande disponibilità, ma anche per la pazienza con cui si sono confrontati con noi su temi che talvolta potevano sembrare anche un po' esotici, ma che in realtà rivestono grande importanza per le popolazioni che vivono nei nostri territori ai confini con la Francia, l'Austria e la Svizzera, le quali hanno esigenze e problemi spesso molto diversi

questo sarà molto probabilmente il mio ultimo intervento in quest'Aula. Devo dire che, delle sei legislature che ho fatto, quest'ultima in Senato è stata senz'altro per me la più bella per l'ottimo clima clima di collaborazione che si è creato non solo con il Governo, ma anche con i colleghi Capigruppo e i funzionari del Senato. Ho trovato sempre un grande rispetto per la nostra diversità di lingua, In questo - devo ammetterlo - l'Italia e la sua classe dirigente si sono sempre contraddistinti positivamente rispetto ad altri Paesi, come la Spagna, la Francia o la Grecia, che hanno avuto un atteggiamento molto

se non avessimo avuto personaggi come Aldo Moro, Giulio Andreotti, Giorgio Napolitano, Alcide Berloffa e Silvius Magnago? Molto probabilmente oggi saremmo ancora una Provincia povera, afflitta da conflitti etnici, in forte contrapposizione

Settanta, grazie all'autonomia speciale, il nostro territorio si è evoluto, tanto da vantare oggi la piena occupazione, il PIL *pro capite* più alto delle Province italiane e con un residuo fiscale di 2.300 euro, rientrando così nel novero delle poche Regioni italiane in attivo, dietro solo alla Lombardia, all'Emilia-Romagna e al Veneto nella contribuzione verso le casse dello Stato. Paghiamo molto più di altre Regioni del Paese che sono in*deficit*. Colgo, quindi, l'occasione per ringraziare il Governo e questo Parlamento per la lungimiranza e l'oculatezza delle scelte effettuate. Sono sicuro che, nello spirito che ha sempre animato le forze politiche

Signor Presidente, dopo il passaggio alla Camera non resta che confermare il giudizio negativo del Gruppo Articolo 1 - MDP - Liberi e Uguali su una manovra di bilancio che ripete stancamente ricette cui manca una visione complessiva; ricette che si sono già mostrate inadeguate, sbagliate, non in grado di garantire al nostro Paese una crescita economica degna di questo nome, che sia, cioè, guidata dagli investimenti e che sia sostenibile dal punto di vista ambientale e sociale. Particolarmente dolente sotto questo profilo per noi è il capitolo della sanità, che resta ampiamente sottofinanziata e con riferimento alla quale da tempo denunciamo il rischio che si comprometta definitivamente un servizio universale, confinando la salute a un privilegio per pochi. Particolarmente grave sotto questo profilo è la farsa della mancata abolizione del superticket. Visto il poco tempo a disposizione, voglio sottolineare, per quanto riguarda il merito, il tema della legalità, un tema per noi imprescindibile. Sono due gli elementi peggiorativi, cui ci siamoopposti con tutte le nostre forze, che questo disegno di legge introduce in materia di certificazione antimafia, smentendo scelte compiute da queste Camere solo pochi mesi fa con la riforma del codice antimafia. Per un verso, si esentano da certificazione le imprese agricole che hanno richiesto sussidi all'Unione europea entro il limite di 25.000 euro (e questa è colpa del Senato); per altro verso - e questa è colpa della Camera - si reintroduce una soglia al di sotto della quale i consorzi di società non devono chiedere la certificazione.

voglio stigmatizzare la violazione di ogni regola con l'introduzione affrettata di interi disegni di legge - chiaramente ordinamentali - senza tenere in alcun conto il dibattito che su di essi si era compiuto nelle Commissioni di merito. Vorrei infine sottolineare, ribadendo il voto contrario del mio Gruppo, che il contributo più visibile della Camera a questo provvedimento è stato, purtroppo, l'approvazione di un insieme infinito ed elettoralistico di microinterventi, che rappresentano un'interpretazione povera, vorrei dire misera, di cosa voglia dire per un parlamentare interessarsi del proprio territorio. Ma di questo tema - lo sappiamo - in questi giorni si parla spesso a sproposito.

Detto questo, il vero problema è che due anni fa si è modificata la legge di contabilità, che ha portato a questa nuova legge di bilancio.

bene. Questa legge di contabilità, quindi, doveva portare alla soluzione di tutti i problemi. Invece, mi pare di capire che nessuna modifica legislativa può portare alla soluzione dei problemi perché esiste sempre, purtroppo (o per fortuna, ma dipende dalle persone), la discrezionalità personale di chi poi va a applicare queste leggi, compresa la legge di contabilità. Anche qui, un esempio su tutti. Nella legge di bilancio di quest'anno, nonostante non si possano fare norme prive di effetti finanziari, alla Camera è stata modificata la legge elettorale all'interno della legge di bilancio, che è una cosa da

Quindi, non è cambiando le regole che si risolvono i problemi relativi ai buchi di bilancio. Purtroppo, i problemi si risolvono cambiando la struttura mentale delle persone che hanno l'onore di mettere le mani sul bilancio dello Stato. Chi va a gestire il bilancio dello Stato deve pensare al bene del Paese e al bene dei cittadini. Non deve trasformare questo onore che ha, qui in quest'Aula, in una

Ovviamente, noi voteremo «no» a questa legge di bilancio, come abbiamo sempre votato «no» alle altre leggi di bilancio. Ma l'augurio è davvero che chi in futuro prenderà in mano questo Paese - chiunque sia

che sarà difficilmente sanabile, perché equivale praticamente a una legge di bilancio all'anno solo di clausole. Colgo l'occasione per fare a tutti gli auguri, ma soprattutto per ringraziare chi ci ha supportato e seguito in questi anni,

una politica economica fallimentare, fatta di debito (anche questa manovra è fatta a debito), di una politica finanziaria che lascia un Paese sepolto dal *deficit*, che renderà davvero difficile il compito di chi verrà dopo, anche grazie alle clausole di salvaguardia di 50 miliardi che ci lascia questo Governo.

stati cinque anni particolarmente difficili, con una politica economica caratterizzata dai *bonus* e dal «tassa e spendi». Questa finanziaria è esondata alla Camera e neanche il povero vice ministero Morando è riuscito a ricondurla in un argine normale. Tanti anni di provvedimenti annunciati, ma mai adeguatamente finanziati. Il lavoro è un tema che è passato più sulla bocca dei parlamentari che nei fatti; il lavoro non si crea con una legge, ma aiutando le imprese a fare lavoro. Sono stati cinque anni nei quali abbiamo assistito

di un loro diritto. Cinque anni di moltissima demagogia che non è servita certo a fare crescere il Paese; cinque anni in cui abbiamo perso il treno congiunturale che fortunatamente ci si era presentato, con Draghi che ci ha aiutato, il prezzo del petrolio che per tanto tempo è stato veramente basso, il rapporto con il dollaro che ci ha aiutato fin quando abbiamo potuto avvantaggiarcene. Ma non siamo stati in grado di riprendere la crescita e siamo fanalino di coda in un'Europa che sta andando molto più veloce di noi. Un'Europa in cui non siamo stati in grado di incidere minimamente in questi cinque anni; politiche dei migranti spesso incoerenti; abbiamo perso la grande occasione di EMA, nonostante avessimo il migliore *dossier* non siamo stati assolutamente incisivi in tutti questi anni di politica che abbiamo vissuto al margine. Quindi, è sicuramente un bilancio negativo, ed è per questo che Forza Italia, dopo questi cinque anni di coerente politica contraria anche alle politiche economiche del Governo, si presenta serena agli elettori, davvero serena, perché saprà intercettare il consenso che il presidente Berlusconi sarà in grado di riportare in campagna elettorale. Il centrodestra non è stato demolito da questi cinque anni, ma ha trovato proprio nella coerenza la forza di rinascere e di proporre ora una vera alternativa a questo Governo disastroso e alla sinistra. Per questo motivo, signor Presidente, vorrei ringraziare, a nome del presidente Romani, tutte le persone che ci hanno consentito di fare questi anni di legislatura, gli uffici e i nostri collaboratori.

Signor Presidente, senatrici e senatori, il disegno di legge che ci apprestiamo a votare è l'atto conclusivo del ciclo di bilancio per l'anno in corso e l'ultima manovra della legislatura in corso. Il provvedimento si inserisce pienamente nel solco degli interventi di politica economica e di finanza pubblica adottati sin dall'avvio della legislatura che hanno consentito al nostro Paese di uscire da una situazione di grave crisi economica e finanziaria, fra le più gravi registrate dalla nascita della Repubblica, e di agganciare la fase di ripresa in atto nel contesto internazionale. Ora siamo di fronte ad un quadro completamente diverso rispetto a quello di inizio legislatura e nelle condizioni di guardare al futuro con buone prospettive di migliorare le condizioni di benessere economico e sociale dei cittadini: numerosi dati macroeconomici recentemente diffusi dall'ISTAT ci illustrano questa inversione di rotta. quindi noi a dirlo, ma dati significativi presentano un Paese che c'era prima e uno che c'è ora, sul prodotto interno lordo, sul numero degli occupati, sui consumi finali, sugli investimenti, sull'*export*. Analogamente, il quadro di finanza pubblica presente una situazione di forte miglioramento rispetto alla situazione di inizio legislatura. Il *deficit* pubblico è sotto controllo, l'avanzo primario è fra i migliori registrati nell'ambito dei Paesi membri dell'Unione europea; il debito pubblico, per la prima volta dopo diversi anni di crescita inarrestabile, ha invertito il proprio percorso e nei prossimi anni tornerà a scendere ad un ritmo sostenuto. Lasciamo un Paese con i conti in ordine.

Possiamo essere orgogliosi di questa legislatura, possiamo esserlo tutti, maggioranza e opposizione. Abbiamo lavorato tanto, ciascuno nel proprio ruolo, e lasciamo un Paese davvero diverso da quello che gli italiani ci hanno affidato il 15 marzo 2013. È stata anche una grande stagione dei diritti, che ha toccato nell'intimo la vita di tante donne e di tanti uomini. Sono emozionata di svolgere quest'ultimo intervento in Assemblea e ringrazio il senatore Zanda di avermi concesso questo privilegio. Ringrazio il PD, i Gruppi di maggioranza e il Governo per il risultato conseguito in questi anni e in particolare per la chiusura di questo bilancio non facile, ma che mette in sicurezza la finanza pubblica in un periodo delicato, come sarà il primo semestre del 2018. Ho un augurio: che il futuro del nostro Paese sia lieve, noi abbiamo cercato di lavorare in questa direzione. Possiamo votare con orgoglio questa fiducia e dichiaro pertanto il voto favorevole del Gruppo Partito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

senatore Dalla Zuanna. Ricordo a tutti che dopo il voto di fiducia ci saranno le votazioni sugli emendamenti e gli articoli e a seguire anche i voti per i giudici amministrativi,

Spilabotte, Sposetti, Stefano,

votazione nominale con appello dell'articolo 1 del disegno di legge n. 2960-B, nel testo approvato dalla Camera dei deputati, sul quale il Governo ha posto la questione di fiducia:

del disegno di legge. Passiamo all'esame dei restanti articoli del disegno di legge. Con l'approvazione dei singoli articoli si intendono approvate anche le tabelle, i i quadri generali, gli allegati e gli elenchi richiamati dagli articoli stessi e riportati negli stampati del disegno di legge. Passiamo alla votazione

Dichiaro aperta la votazione

tutti quanti i senatori. Ringrazio inoltre il segretario generale, dottoressa Serafin, i Vice Segretari generali e tutti i dipendenti che mi hanno aiutato a svolgere come ho potuto la mia funzione di Presidente. Avrei voluto salutare anche tutti i dipendenti con una cerimonia singola proprio perché era la fine della legislatura, ma i frenetici lavori parlamentari degli ultimi giorni non mi hanno consentito di farlo in uno specifico momento come avrei voluto, un saluto a tutti i dipendenti in maniera particolare. si leva in piedi)*. Un saluto anche ai componenti del Governo che sono qui presenti e che hanno collaborato nella nostra funzione.

della Giustizia amministrativa, della Corte dei conti e della Giustizia tributaria. Intervengo ancora con più convinzione in seguito al fatto che questa stessa votazione alla Camera dei deputati non è stata effettuata nella giornata di ieri, come invece era previsto. Non si è effettuata perché non c'era condivisione sulle liste, così come dovrebbe essere, né fra i Gruppi parlamentari, né fra Camera e Senato. Ebbene, Presidente, noi riteniamo questi organi fondamentali soprattutto perché particolarmente vicini ai cittadini. Le chiedo quindi di bloccare, fermare la militarizzazione politica su queste nomine, perché non possiamo permettere che a fine legislatura i partiti possano spartirsi le poltrone attribuendole a politici di professione, militarizzando appunto tali ruoli e non lasciando che a ricoprirli siano soggetti di elevata competenza e professionalità. Si tratta, evidentemente, di organi delicati di autogoverno di magistrature specializzate. Risulta dunque imprescindibile un profilo soggettivo di notoria indipendenza, di autorevolezza morale, di imparzialità e di elevata competenza. Attingere dal bacino dei politici pare del tutto sconveniente, gravemente inopportuno e si rischia, oltretutto, di minare la funzionalità e la legittimità dei predetti organi. È necessario rispettare il senso formale e sostanziale delle norme che disciplinano l'elezione di tali Consigli di Presidenza ed ed è quindi aberrante trasformarli in parcheggi d'oro per parlamentari in scadenza. Noi abbiamo adottato un metodo ed è quello di aver individuato i profili migliori,

io credo che sarebbe opportuno un suo autorevole intervento, anche alla luce di quanto da lei stesso più volte ribadito in quest'Aula e fuori da quest'Aula in forza della sua funzione istituzionale di garante. Piuttosto che questo scempio, sarebbe quantomeno opportuno rinviare la votazione soltanto in presenza di liste dignitose, con soggetti idonei ai ruoli, con profili pienamente rispondenti alle delicatissime mansioni da svolgere e di certo in presenza di una piena condivisione da parte di tutti i Gruppi che non c'è

perché tante cose abbiamo fatto noi che l'altra Camera non è riuscita a fare e questo non ci può assolutamente bloccare, quindi questa non può essere una motivazione. *(Applausi dal Gruppo

prego.

sui nomi (come tutti i colleghi senatori), cognizione di causa, perché per deliberare, come ha ricordato lei oggi, bisogna conoscere. Noi conosciamo due colleghi, che sono qui presenti

Signor Presidente, desidero annunciare che anche il mio Gruppo non parteciperà al voto, perché la ripartizione tra Gruppi che emerge da questo insieme di nomi che ci è stato dato *in camera caritatis* dimostra che c'è stato un accordo fra Gruppi che hanno i numeri per sostenere la loro propria proposta,

sulla base delle designazioni pervenute dai Gruppi: - professor Saverio Ruperto - avvocato Gianluca Susta. Ricordo che, in base alla citata disposizione di legge, i due candidati saranno proclamati eletti se la lista otterrà la maggioranza assoluta dei voti dei componenti l'Assemblea, cioè 161 voti. I senatori favorevoli alla lista proposta voteranno sì; i senatori contrari voteranno no; i senatori che intendono astenersi si comporteranno di conseguenza.

Evidentemente non si è raggiunto il *quorum* di 161. Procediamo alla votazione per l'elezione di due componenti del Consiglio di Presidenza della Corte dei conti, ai sensi dell'articolo 7, comma 1, lettera *d)*, della legge 27 aprile 1982, n. 186, e dell'articolo 18, comma 3, della legge 21 luglio 2000, n. 205. Tale votazione avverrà a scrutinio segreto, ai sensi dell'articolo 25, comma 3, del Regolamento, sulla seguente lista compilata sulla base delle designazioni pervenute dai Gruppi: - avvocato Ciro Falanga - professor Maurizio Leo. Ricordo che, in base alle citate disposizioni di legge, i due candidati saranno proclamati eletti se la lista posta in votazione otterrà la maggioranza assoluta dei voti

sulla seguente lista compilata sulla base delle designazioni pervenute dai Gruppi: - professor Antonio Carullo - avvocato Gianfranco Schietroma. Ricordo che, in base alla citata disposizione di legge, i due candidati saranno proclamati eletti se la lista posta in votazione otterrà la maggioranza assoluta dei voti dei componenti l'Assemblea, cioè 161 voti.

sulla questione se il Senato debba promuovere conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato innanzi alla Corte costituzionale con riguardo agli atti posti in essere nell'ambito del procedimento penale pendente presso il tribunale di Verona

che, come lei ha anticipato, chiede di sollevare il conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato, perché deve essere chiarito se l'esercizio della funzione legislativa sia o no sindacabile giurisdizionalmente, trattandosi in questo caso di un procedimento nel quale si contesta la corruzione per la presentazione e il sostegno di un emendamento. come dice la Corte costituzionale, siamo nel punto centrale della funzione parlamentare; siamo allo snodo del rapporto tra politica, potere legislativo e potere giudiziario sul punto del chiarimento dei dei limiti dell'autonomia delle Camere e dei parlamentari, autonomia sancita dall'articolo 68, primo comma, dall'articolo 64 e dall'articolo 72 della Costituzione.

alla sua elezione all'Assemblea regionale siciliana. Trattandosi di un caso d'incompatibilità ai sensi dell'articolo 122 della Costituzione, il Senato non può che prenderne atto.

simultaneo della proposta della Giunta delle elezioni e delle immunità parlamentari di promuovere conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato dinanzi alla Corte costituzionale, con riguardo agli atti posti in essere nell'ambito del procedimento penale pendente presso il tribunale di Verona anche nei confronti della senatrice Bonfrisco.

La Presidenza si intende pertanto autorizzata a dare mandato a uno o più avvocati del libero foro.

Presidente, comprende anche lei che non si riesce neppure ad argomentare con questo caos. *(Commenti di solito c'è anche più rumore di fondo. CANDIANI *(LN-Aut)*. Senza dubbio, capisco che questo poi sia un argomento a cui lei tiene particolarmente. È stato presentato un testo scritto, al quale mi rimetto, che illustra la questione pregiudiziale che chiediamo venga posta in votazione.

«*Ius soli*, bene lo *stop*, il Paese è già lacerato». «Il segretario di Stato Vaticano: legge controversa, serve un consenso

e mentre in Parlamento echeggiavano gli ultimi accesi appelli pro *ius soli*, il cardinal Pietro Parolin, al Ceis per la messa natalizia commentava con una buona dose di concretezza lo *stop* di una delle leggi più care al mondo cattolico. Deluso? Si pensava potesse essere approvata ma ci sono state troppe reazioni negative. È apparsa come una legge controversa suscitando risposte diverse da parte di tanti settori dell'opinione pubblica e della gente. Davanti a un quadro del genere occorre avere il tempo necessario per maturare, per convincere, in modo tale che il passo successivo lo si possa fare ma con il maggior consenso possibile». «Penso che sia meglio che queste cose abbiano lo spazio temporale per maturare a livello di coscienza e mentalità, affinché non siano fonte di conflitto e di lacerazione dentro il Paese».

A me sconcerta il giochino del chi tiene in mano il fiammifero e alla fine si scotta, perché mai avremmo dovuto essere in questo momento a discutere su un argomento del genere. Diversamente, diventa veramente una presa in giro e le parole di monsignor Parolin mi sembra dicano esattamente il contrario. Tutti sappiamo che il provvedimento non andrà mai in porto, perché ho presentato 50.000 emendamenti non ho sentito richieste di fiducia da parte del Governo, né ho sentito autorizzare la fiducia. Pertanto, che la sinistra rispetto alla sinistra estrema, rispetto alla sinistra di mezzo facciano a gara per scaricare l'un l'altra la responsabilità, per me è un segno di irresponsabilità perché giusta o sbagliata che sia questa legge, essa coinvolge una montagna di persone.

le chiedo di verificare la presenza del numero legale.

Conferenza dei Capigruppo e il voto che si è verificato qui, in quest'Aula, in cui noi abbiamo fatto l'ultimo disperato tentativo di inserire il disegno di legge sulla cittadinanza

brutta pagina, un'ipocrisia sulla pelle di tanti ragazzi e ragazze, di circa un milione di persone, uomini, donne e bambini che aspettavano questa legge.

brutta, che avrà delle conseguenze, perché le conseguenze già ci sono, nel nostro Paese. Dispiace che il mio ultimo intervento in quest'Aula debba essere volto a stigmatizzare, ancora una volta,

Signor Presidente, intervengo solo per rimandare al mittente le ingiustificate accuse del senatore Calderoli per quanto riguarda il mio Gruppo. Da quando questo Gruppo si è costituito, ha chiesto

questo provvedimento. Sappiamo benissimo che non ci sono state le condizioni per farlo prima, a causa delle grandi spaccature all'interno dei Gruppi di sinistra ritengo che davvero non sia il momento per il Paese, perché questo provvedimento creerà certamente forti tensioni sociali. Invito i Gruppi della sinistra

Presidente, senatrici e senatori, trovo assai interessante, ma anche un filo bizzarro, del senatore Calderoli, a favore della pregiudiziale di costituzionalità, sia stato interamente condizionato da un'impostazione schiettamente clericale, che faceva, cioè, riferimento alle considerazioni di una voce altamente autorevole e significativa delle gerarchie cattoliche, voce che non è certo quella che deve organizzare, determinare e orientare il dibattito nell'Aula del Senato della Repubblica. A questa impostazione schiettamente clericale poi si è aggiunto un tipo di considerazione di natura agonistica, secondo il paradigma della lotta greco‑romana, che fa riferimento a quei 50.000 emendamenti, branditi come un arma impropria. Ebbene, penso che questa impostazione sia davvero profondamente errata. Noi siamo in presenza di una grandissima questione che, giustamente, in molti considerano trattata con colpevole ritardo a causa degli errori fatti da molte parti politiche, compresa quella alla quale io appartengo. Non dobbiamo, però, dimenticare il merito della questione. Ciò che domina nell'attuale nell'attuale normativa sulla cittadinanza è il cosiddetto *ius sanguinis*, che è una impostazione che, come sanno coloro che questa materia hanno studiato, risente di una cultura di tipo elementare, primitiva, vorrei dire barbarica, fondata appunto sullo *ius sanguinis* e, quindi, sull'idea di una *enclave* chiusa, autoreferenziale, destinata fatalmente fatalmente a un inevitabile esaurimento e inaridimento. All'opposto, lo *ius soli* è parte integrante della nostra civiltà giuridica. conseguenza di una cultura e di una tradizione che ha i suoi fondamenti nella tradizione greca e in quella latina e che si fonda, all'opposto dello *ius sanguinis*, su una idea di cittadinanza costituita intorno alla coesione sociale, alla condivisione di diritti e doveri, alla profondità del legame sociale, alla reciprocità, cioè a una idea tutta evolutiva legata, appunto, alla crescita del diritto contemporaneo. Noi abbiamo, di fronte a noi, questa contrapposizione netta tra due impostazioni: uno *ius sanguinis* di origine e connotati profondamente premoderni e uno *ius soli* che corrisponde alle esigenze, alle trasformazioni profonde, alle volontà di quelli che sono gli attuali cambiamenti a livello mondiale e nella nostra area. Siccome abbiamo tempi ridotti, mi

intervengo per esprimere il voto contrario alle questioni pregiudiziali di costituzionalità poste e per sostenere la posizione dei socialisti presenti in quest'Aula sulla volontà di dare attuazione alla modifica della legge sulla cittadinanza, che non è un riconoscimento automatico del diritto di cittadinanza, ma è un percorso giusto e legittimo per dare a coloro che nascono

che non è soltanto comunità di sangue, ma è comunità d'impegno, di cultura, di coinvolgimento e anche di contributo civico all'attività del Paese. Noi oggi rimediamo a una ingiustizia che da troppi anni permane nel nostro Paese. Qui non si tratta di mischiare capra e cavoli: immigrazione, pericoli e terrorismo. Tutto questo armamentario, francamente, è scarsamente democratico e razionale rispetto a una problematica che deve vedere accolti nella nostra comunità nostra comunità questi cittadini, che sono nati, che sono immigrati in Italia e che danno il loro contributo a questo Paese. Esprimo quindi la volontà di proseguire con la votazione del contenuto di questa proposta di legge. Signor Presidente, per un problema di coscienza voglio anch'io lasciare agli atti del Senato che - lo dissi la prima volta quindici anni fa, da Presidente della Camera - sono favorevole al provvedimento e voterò contro le pregiudiziali di costituzionalità.

seduta, a volte il Natale arriva ed io auguro veramente un sereno Natale alle vittime del Forteto. Mi mancherà l'attività legislativa e mi mancheranno meno i senatori.